Ricordiamo che l'Italia è uno dei nove Paesi dell'Unione europea a non avere ancora ratificato l'Accordo in esame, mentre gli altri 17 Stati membri dell'Unione europea hanno già provveduto a ciò. Pertanto, la ratifica si pone come urgenza per armonizzare l'ordinamento italiano a quello degli altri Paesi e per fare entrare finalmente in vigore ‑ lo dico almeno sollevato ‑ questo Trattato. Si spera che anche gli altri accordi seguiranno velocemente lo stesso *iter* in tutti i Paesi comunitari. Ebbene, cari colleghi, l'importanza di fare entrare in vigore gli accordi è dettata, *in primis*, da considerazioni economiche. Secondo quanto riportato nella relazione introduttiva, i costi stimati del programma satellitare si attestano sui 3,2 miliardi di euro. La Commissione europea conta di reperirne due terzi dal settore privato e la restante quota dagli Stati membri. Si deve perciò considerare che l'Unione europea ha assunto impegni per un ulteriore finanziamento del sistema satellitare cui farà fronte con mezzi propri. Voglio appunto sottolineare il Trattato non prevede oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché l'Accordo sarà finanziato con fondi del programma Galileo, che riceve già il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale europea. Tuttavia, è dal mercato che l'Accordo prevede di ricevere i maggiori fondi dato che si progetta l'ingresso di capitali privati in considerazione del fatto che, a breve termine, il sistema dovrebbe generare utili.

la ratifica, che permetterà l'entrata in vigore del Trattato, e la *partnership* con gli altri Paesi extraeuropei, che permetterà un'estensione dello stesso, sono fondamentali per conseguire una celere capitalizzazione privata del sistema, una rendita propria dello stesso e, pertanto, anche la possibilità di reinvestire i finanziamenti dell'Agenzia spaziale italiana tramite l'Agenzia spaziale europea in altri settori di ricerca e di sviluppo. cari colleghi, vediamo che la politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere a disposizione dell'Unione europea due sistemi di navigazione satellitare GNSS (**Global**

in Commissione dai colleghi, è esclusivamente civile. Vorrei poi fare una riflessione specifica sull'Ucraina. Questo Paese è un *partner* diverso e davvero strategico, poiché *leader* mondiale della progettazione e produzione di sistemi di veicoli di lancio e componenti dei sistemi GNSS, e inoltre - come si evince dalla relazione - è l'ottavo è l'ottavo Paese su scala mondiale in materia di programmi spaziali. Non solo si compie la scelta di allargare l'attività del sistema satellitare, dunque, ma anche di allargarla a *partner* competitivi e competenti.

questo non si limita alla facilitazione e al miglioramento della cooperazione in riferimento al sistema satellitare civile, ma le parti possono estendere i settori di cooperazione, attraverso un accordo separato successivo, al comma 2, a tutta una serie di attività connesse al sistema Galileo. Si tratta, quindi, essenzialmente di tecnologie e di beni sensibili nel territorio della Comunità europea, a restrizioni all'esportazione, in relazione alla non proliferazione degli armamenti, nonché di diversi aspetti relativi alla sicurezza del sistema, come gli scambi di informazioni classificate. Considerando dunque l'Accordo come prodromico ad una cooperazione in campo scientifico e spaziale sempre più ampia con l'Ucraina, non posso che sottolineare l'importanza di questa ratifica e augurarmi la velocizzazione delle altre ratifiche, il cui *iter* in questo momento sta andando avanti anche grazie al lavoro che si compie nella nostra Commissione.

inoltre al Governo di interessarsi in sede europea circa l'effettivo completamento del programma Galileo e la limitazione, se non l'eliminazione, dei costi aggiuntivi per il lancio e il posizionamento in orbita dei 30 satelliti previsti. Questa iniziativa è senz'altro ammirevole e assai rilevante sotto il profilo strategico e finanziario, in quanto svolgerà anche importanti funzioni relative ad operazioni di sicurezza, interventi per aiuti umanitari, evacuazione di popolazioni in caso di sciagure, e missioni di pace in contesti di crisi. Ci saranno inoltre applicazioni nel campo dell'osservazione ambientale e del monitoraggio dei movimenti geologici.

Come per gli altri accordi, i meriti di atti bilaterali come questo si trovano nell'apporto che forniscono per chiarire alcuni concetti giuridici, come l'ambito successivo e quello oggettivo di applicazione, ossia persone residenti, da un lato, e redditi e patrimonio, dall'altro, in modo da rendere più semplice l'applicazione burocratica, nel concreto le procedure per il pagamento dei tributi delle operazioni transfrontaliere. Questo è acuito dal fatto che tutti gli accordi ratificati finora sono costruiti sulla base del modello OCSE. In secondo luogo, hanno carattere di equità contributiva, poiché permettono di distribuire equamente il reddito da imposizione fiscale tra le parti contraenti. L'Italia e la Slovenia sono vicine geograficamente; lo sono a livello culturale lo sono a livello comunitario, in quanto condividono il programma di cooperazione transfrontaliera per gli anni 2007‑2013. Sono anche vicine economicamente, se si considera che l'Italia è il secondo *partner* della Slovenia dopo la Germania e che l'interscambio 2007 è pari a 6.500 milioni di euro (di cui l'*export* verso la Slovenia per 4.000 milioni di euro e l'*import* dalla Slovenia per 2.500 milioni di euro)

una più profonda cooperazione economica con un *partner* in crescita sia fondamentale per l'Italia e per la sua economia, visto lo stato in cui versa questo ultimo periodo.

il provvedimento in titolo è d'iniziativa governativa e reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, L'Accordo si inquadra nel novero delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia. Quanto ai contenuti, esso si applica all'imposizione sui redditi, essendo stata reciprocamente esclusa la tassazione del patrimonio. La struttura ricalca il modello degli accordi di specie riconosciuti internazionalmente ed elaborati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Questo mi esula dall'entrare nel merito delle questioni e mi consente di rimettermi

senatore Pedica.

del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Essa assoggetta a distinti regimi di protezione le categorie di beni tutelati, prevedendone la protezione da parte delle forze armate nazionali degli Stati contraenti per evitare il saccheggio e la sottrazione. Quanto al contenuto del disegno di legge abbiamo delle disposizioni di adattamento della nostra normativa interna che derivano dalla necessità di individuare le misure propedeutiche di salvaguardia dei beni culturali, con riferimento alle disposizioni già vigenti in materia di tutela di beni culturali e del paesaggio. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno riguardato in particolare due articoli, il 6 e il 15, che contengono disposizioni in materia penale e che introducono le fattispecie dei reati militari in danno di beni culturali previsti dal Protocollo. L'articolo 6, in particolare, individua nei conflitti armati e nelle missioni internazionali l'ambito temporale di applicazione della disciplina penale e precisa l'estensione in relazione sia all'autore, che al luogo del commesso reato. Questo è il contenuto della Convenzione che propongo all'Assemblea di approvare. PRESIDENTE.

alla protezione del patrimonio culturale nel caso di conflitti armati, è stata originata dalla consapevolezza delle irreparabili distruzioni di patrimoni culturali causate dal perdurare negli anni di tragici conflitti. Data, appunto, la matrice storica, il primo Protocollo alla Convenzione è quello relativo alla protezione del patrimonio culturale in tempo di occupazione. Quindi, per completare il quadro normativo e attualizzarlo, nel 1999, si è provveduto a realizzare il secondo Protocollo alla Convenzione, ossia quello che oggi ci si propone di ratificare, unitamente a norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale. Questo secondo Protocollo prevede un regime di protezione dei beni artistici che è ulteriore rispetto agli altri due già determinati, e cioè la protezione rafforzata. La protezione rafforzata si realizza tramite la redazione di una lista internazionale, compilata sotto il controllo di un apposito comitato intergovernativo, che raccoglie tutti quei beni culturali (anche quelli di casa nostra e vorrei continuare a far riflettere chi non interviene),

Il comitato intergovernativo valuta le proposte formulate da ciascuno Stato contraente e delibera a maggioranza qualificata l'inclusione nella lista. L'elenco è poi reso noto a tutti gli Stati aderenti, all'UNESCO ed all'ONU, e quindi ha valenza internazionale.

L'esame in seconda lettura è pertanto limitato alle parti oggetto di modifica. L'altro ramo del Parlamento ha offerto il proprio contributo alla sua elaborazione, introducendo modifiche in materia di diritto penale sostanziale (in particolare, una diversa qualificazione di alcuni speciali reati militari e di alcune circostanze aggravanti e relativo profilo sanzionatorio). Le pene previste, cari colleghi, non sono certo di lieve entità, come è giusto che sia, in quanto all'articolo 10 si dispone che: "Chiunque illecitamente distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile un bene culturale protetto dalla Convenzione, è punito con la reclusione da due a otto anni." Di questo, l'Italia dei Valori fa anche un vanto, avendo portato a compimento una battaglia per indurre queste persone a non delinquere appunto la pena ad un inasprimento che avrei preferito maggiore. Vorrei sottolineare che alla Camera si è modificata anche la copertura finanziaria prevista dall'articolo 16 e cioè si è previsto di far fronte alla spesa, peraltro assai limitata, di 8.980 euro per l'anno 2008 e ‑ qui invito i colleghi a riflettere e il Governo a rispondermi di 4.890 euro per il 2009 e di euro 8.980 a decorrere dall'anno 2010 ‑ non sono milioni, ma migliaia di euro mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma Fondi di riserva del Ministero dell'economia e delle finanze. Tra le modifiche si deve sottolineare anche che, in relazione al cittadino straniero, si è stabilita l'applicazione della Convenzione a tutti i reati previsti dal disegno di legge, anziché solo ad alcuni, a condizione che lo straniero si trovi nel territorio dello Stato italiano. Come Come dicevo in apertura del mio intervento, e come ha sottolineato il relatore, merita una riflessione il fatto che normalmente la ratifica di accordi internazionali avviene con disegni di legge di due articoli soli, mentre nel disegno di legge n. 1073 si regolano molti più aspetti perché si deve modificare la nostra normativa interna. La normativa nazionale della materia riguardante i beni culturali è contenuta nel citato codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, il quale, pur contenendo una sua disciplina sanzionatoria penale, non contempla alcune fattispecie penali previste dagli articoli 15 e 21 del Protocollo. In generale, nel codice nel codice di beni culturali assume rilievo non l'offesa al bene in sé, ma l'intralcio alla funzione amministrativa di controllo esercitata dagli organi competenti sulle attività concernenti il bene culturale. Si evidenzia, infine, una categoria particolare di indiretti destinatari del Protocollo, ossia i comandanti militari, cui compete il rispetto degli obblighi sanciti in merito alla conduzione delle operazioni militari offensive e difensive, nonché dei divieti e limiti che incombono sulle forze occupanti nel territorio di Stati esteri durante le operazioni di mantenimento della pace. Tuttavia, colleghi, colleghi, devo far presente come l'indirizzo generale del Protocollo è già adottato dalle Forze armate italiane, attualmente impegnate in importantissime missioni all'estero, alle quali vorrei porgere un saluto e un ringraziamento per il lavoro a tutela della pace e della sicurezza.

il Protocollo aggiuntivo della Convenzione dell'Aja del 1954 è entrato in vigore sul piano internazionale nel 2004 e l'Italia ha assicurato la partecipazione dei propri rappresentanti agli organismi intergovernativi soltanto come osservatore. pertanto, la ratifica dell'accordo internazionale perché possa partecipare come membro ai prossimi incontri di questo anno fissati a Parigi.

la causa delle ratifiche che abbiamo portato al voto. Credo che l'Italia dei Valori sia soddisfatta di aver contribuito a questa ratifica, mettendoci

Premetto subito che il mio Gruppo, l'Italia dei Valori, considera importante ratificare questo protocollo allegato alla Convenzione dell'Aja del 1954, innanzi tutto per le ragioni storiche che ho precedentemente illustrato.

ricettazione di manufatti archeologici e storico-artistici da parte di trafficanti internazionali, militari, giornalisti e rappresentanti di organizzazioni governative e non governative. Abbiamo vissuto e viviamo nel nostro Paese questi continui furti e saccheggi:

Quindi, a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori, in ragione degli alti fini di questo Protocollo, nonché del positivo accoglimento del contributo del Gruppo della Camera,

Onorevoli colleghi, è con commozione profonda che ricordo oggi all'Assemblea la scomparsa, avvenuta a Roma nella notte tra venerdì e sabato, del collega senatore Ugo Martinat. Nato a Settimo Torinese nel 1942, fu politico di grande esperienza, maturata in anni di lavoro quotidiano dedicato in primo luogo ai problemi del suo territorio e dei suoi concittadini; verso di loro sentiva con forza - nei diversi incarichi ricoperti - il dovere di esercitare il proprio mandato con impegno e passione, rappresentandone sempre con decisione le aspirazioni e le richieste. Dedicatosi in giovane età alla vita politica locale in seno alle organizzazioni giovanili del Movimento Sociale Italiano, venne presto conosciuto ed apprezzato, iniziò a partecipare alla vita del partito anche in ambito nazionale, senza perdere però mai il contatto con la politica torinese, della quale rimase protagonista di primo piano. Di questa sua passione, di questo suo impegno concreto nel fare, amici ed avversari sempre gli diedero atto, riconoscendogli una non comune capacità di affrontare i problemi per risolverli, e non solo per discuterne. Nel 1973 fu eletto nel Comitato centrale del partito, e dal 1979 entrò a far parte della Direzione nazionale. Nello stesso anno, al principio dell'VIII Legislatura, venne eletto per la prima volta deputato, all'età di trentasei Il suo impegno nell'esercizio del mandato parlamentare, rigoroso e attento alle esigenze degli elettori, gli valse, grazie al sostegno costante del corpo elettorale, la conferma nell'ufficio di deputato per tutte le successive Legislature, fino al 2006. Nel corso della XIII Legislatura, Ugo Martinat fu chiamato a ricoprire la delicata e prestigiosa funzione di Questore della Camera dei deputati. Come di consueto, anche questo difficile incarico fu svolto con disciplina e serietà, guadagnando l'apprezzamento sincero di tutti i colleghi. Nella successiva XIV Legislatura, con la costituzione del II Governo Berlusconi, fu nominato Vice Ministro per le infrastrutture e i trasporti, incarico che mantenne anche all'interno del successivo Esecutivo, sino al termine della Legislatura. Nelle elezioni del 2006, terminata l'esperienza di governo, venne eletto senatore per la Regione Piemonte. Nel biennio della XV Legislatura si distinse per un'attività politica e parlamentare condotta con grande vigore, ma sempre nella correttezza e nel rispetto scrupoloso degli uomini e delle procedure. Nel 2008, rieletto senatore, fu chiamato nuovamente a far parte dell'Esecutivo, ricoprendo l'incarico di Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. All'esercizio dell'attività di governo nella quale lo sforzo di contribuire alla salvaguardia e allo sviluppo del nostro sistema produttivo diventava ogni giorno più necessario e più arduo, nel quadro di una difficile congiuntura economica Ugo Martinat ha saputo affiancare, nell'ultimo periodo della sua esistenza, delicati incarichi direttivi all'interno delle strutture piemontesi del suo partito, Alleanza Nazionale, per preparare la costituzione della nuova formazione politica del Popolo della Libertà. Un approdo politico del quale Ugo Martinat non ha potuto vedere - per poche ore - il pieno compimento, nel rammarico di tanti amici, sostenitori e colleghi di partito, e che ha reso, se possibile, ancora più vivi il dolore e la commozione per la sua prematura scomparsa. Lunedì pomeriggio mi sono recato a Torino per portare la partecipazione del Senato della Repubblica alle sue esequie: la grande partecipazione di torinesi e di colleghi parlamentari, anche di parti politiche diverse dalla sua, il clima di viva commozione che si respirava nel Duomo, dimostravano l'affetto e la popolarità di cui godeva quest'uomo, coerente e combattivo, fortemente radicato nei valori e nelle tradizioni della sua parte politica, ma ancora di più immerso nella vita e nella cultura sociale e produttiva del suo territorio. Sono certo di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea nel manifestare ai familiari di Ugo Martinat, ai suoi elettori e al Gruppo parlamentare del Popolo della Libertà il più vivo cordoglio della nostra istituzione ed una sincera partecipazione al loro dolore. Invito, pertanto, tutti i colleghi ad osservare un minuto di raccoglimento.

Colleghi senatori, ci uniamo al cordoglio della Presidenza e ricordiamo la figura di Ugo Martinat: parlamentare di lungo corso, politico serio, capace e preparato Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico di questo Governo. Di lui, in questi giorni, stanno arrivando ricordi toccanti, non solo dalla sua parte politica, ma da tutti gli schieramenti. È vero che la provenienza e gli ideali di Martinat non lasciavano certo spazio a dubbi o a interpretazioni. È stato soprattutto un uomo forte che ha saputo rappresentare per anni lo Stato e le istituzioni con piglio, capacità e pragmatismo, doti che si riconoscono a molti abitanti del suo Piemonte. le stesse doti che lo hanno contraddistinto fin dall'inizio della sua avventura politica. Martinat venne eletto per la prima volta nel 1979 nelle liste del Movimento Sociale Italiano ed in seguito in Alleanza Nazionale. La sua storia politica proveniva da lontano: dai difficili e controversi anni Settanta, quelli degli scontri politici, anche nelle piazze. Nei giorni delle lotte accese, Ugo Martinat lavorò a stretto contatto con Giorgio Almirante e non si risparmiò mai per i suoi ideali. Come sempre in prima linea, perché questo era il suo modo di fare politica, dimostrava grande capacità decisionale, lealtà e schiettezza: qualità che resero Martinat a detta di tutti un protagonista, prima nella sua città, Torino, e poi nel Parlamento nazionale, fino alle responsabilità di Governo. Da tutti i ricordi traspare la grinta e la forza di un uomo che ha sempre difeso strenuamente i suoi ideali. Un deputato di un partito diverso dal suo, ma torinese come lui, ricordandone le qualità umane e politiche, lo ha definito "un combattente indomito, ma leale". Era rispettato, insomma, dai suoi avversari almeno quanto era seguito ed apprezzato dai suoi amici. Ugo Martinat era un politico come ce ne sono sempre meno, appartenente ad una categoria che qualcuno vorrebbe sempre meno presente: è partito dal territorio, dalla base, dal contatto con la gente e a quella sempre si rivolgeva. Nonostante i suoi incarichi si facessero sempre più prestigiosi, non ha perso quell'aderenza con la realtà e con l'elettorato che spesso molti di noi abbandonano colpevolmente col tempo. Per un uomo come lui, schierato decisamente e orgogliosamente a destra, l'appartenenza e il rapporto con lo zoccolo duro del suo elettorato erano tutto. Era gentile e disponibile con chi, come me, spesso condivideva con lui il viaggio verso Torino. In una In una delle sue ultime interviste, avvertiva con preoccupazione i problemi strutturali esistenti nel nostro Paese e in particolare nell'economia italiana. È una triste coincidenza che Ugo sia scomparso proprio nel giorno in cui uno dei suoi progetti, una delle sue più grandi aspirazioni politiche, il Partito della libertà, prendeva il via. La nascita del nuovo soggetto politico, che lui vedeva come un passo decisivo verso l'ambizione antica che si compie, era sempre stata nei suoi pensieri. L'applauso caldo ed appassionato della platea dei delegati, di cui avrebbe senz'altro fatto parte se non avesse dovuto fare i conti con la malattia, vale molto più di qualsiasi frase. senatrice Boldi Signor Presidente, oggi ricordiamo in quest'Aula la figura di Ugo Martinat. Nato a Settimo Torinese nel 1942, dunque piemontese, ha iniziato la sua attività politica nel Movimento Sociale Italiano, caratterizzandosi da subito come un *leader*, ricoprendo incarichi nelle formazioni giovanili e poi nella segreteria del Fronte della Gioventù. Ugo Martinat è stato tra i protagonisti di una stagione politica difficile in una città, Torino, particolarmente colpita e provata negli anni Settanta; una stagione

del genere non si ripresenti mai più nella storia politica italiana. Deputato per la prima volta nel 1979, prima nelle liste del Movimento Sociale Italiano e poi di Alleanza Nazionale, ha seguito tutti i cambiamenti politici del partito fino all'approdo, sicuramente convinto, nel PdL, e penso che sarebbe stato contento di vedere la nascita del del partito che è venuto alla luce la scorsa settimana. L'abbiamo conosciuto come un uomo coraggioso, deciso, leale, molto rispettato

è sempre rimasto legato e anche quando gli impegni nazionali lo portavano lontano, sempre ritornava nella sua città, senza mai dimenticarsi di svolgere attivamente attività politica nella sua città Un uomo che ha vissuto fino in fondo la sua vita, un uomo che lascerà sicuramente una traccia nella storia del Parlamento di cui ha fatto parte sette volte come deputato e poi

voglio testimoniare ai familiari e naturalmente a tutti i dirigenti del PdL, a nome mio personale e del Gruppo Lega Nord, il più sincero sentimento di cordoglio.

Lacultura politica dominante a Torino, anche in forza della storia della città e della Regione, è stata quella del cattolicesimo popolare e democratico, del liberalismo, dell'azionismo, del movimento socialista e comunista. Ugo Martinat rispetto a questo mondo ideale affermò sempre, con una passione indomita e un assoluto convincimento, una posizione politica di minoranza, di controtendenza. Egli fu sempre uomo di minoranza, di controtendenza e talvolta anche uomo contro;

Fu protagonista della vita consiliare comunale torinese. Era un parlamentare, ma anche un consigliere comunale che non mancava di partecipare alle sedute del Consiglio della sua città. Furono memorabili alcune battaglie, come quella che assegnò all'Acqua Marcia di Vincenzo Romagnoli la progettazione del nuovo stadio "Delle Alpi"; si trovò insieme a parte della sinistra a votare contro la proposta di Romiti. Nessuno può non riconoscergli l'impegno grande che lui profuse per la sua città, sia nel facilitare le opere strutturali che poi confluirono nel grande evento olimpico e, più recentemente, per facilitare l'afflusso dei fondi per la metropolitana

all'inizio del 2006, cominciai a fondare il comitato piemontese per il *referendum* elettorale e ci trovammo, cittadini dell'Ulivo, esponenti di varie forze partitiche, professori universitari e lui, per Alleanza ad organizzare il comitato referendario e a raccogliere firme. Fu sempre molto leale e molto discreto; non metteva il cappello della sua forza politica su un'impresa comune.

appoggiato la svolta di Fiuggi, quando parlava a tu per tu pensasse, col sentimento, di poter traghettare tutta intera una storia, tutti interi i simboli, tutta intera una vita

spalle. Voglio quindi associarmi al dolore dei suoi familiari e della sua forza politica; associarmi - così come ha fatto il Partito Democratico nazionale e piemontese ai suoi funerali - nel ricordo di un protagonista di un protagonista che va rammentato nelle sue luci, nelle sue ombre, nella sua verità e nella ricerca intellettuale e morale che ha portato fino in fondo, per un esito di una vicenda nazionale di cui lui è stato un vero protagonista. Grazie, Signor Presidente, onorevoli colleghi, è ovviamente con grandissimo dolore che, a nome di tutto il Gruppo del Popolo della Libertà, ricordo in quest'Aula Ugo Martinat al quale, come molti della mia comunità politica di appartenenza, mi ha legato un rapporto più che decennale; con il quale abbiamo condiviso impegni, traguardi, ansie e battaglie politiche. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare il presidente Schifani, non solo per le parole che prima ha pronunciato in ricordo del senatore Ugo Martinat, ma anche perché con la sua partecipazione, fin dal momento della sua scomparsa avvenuta a Roma sabato mattina, ma poi con la partecipazione calorosa e con grande amicizia alle esequie che sono state celebrate lunedì, ha voluto cogliere non solo l'importanza del ruolo che Ugo Martinat ha svolto nella politica di Torino, del Piemonte, del Parlamento, del Senato e prima ancora della Camera deputati, ma ha colto anche l'importanza che la figura di Ugo Martinat ha avuto per un'intera comunità politica, alla quale ha dedicato un impegno pluridecennale, che anche quest'oggi nell'Aula del Senato vediamo riconosciuto, salutato, indipendentemente dalle appartenenze, indipendentemente dalla diversità di idee che Ugo non ha mai negato, negato, che ha sempre vissuto con grande fierezza e passione, sempre conquistandosi il rispetto di tutti. Nona caso lunedì nel Duomo di Torino erano tanti i gonfaloni di Comuni e di città, non solo Torino, a dimostrazione che Ugo è stato un uomo del territorio, legato a un impegno, sì nazionale, man mano che le sue responsabilità politiche nel Parlamento e nel Governo sono cresciute, ma sempre legato alla sua città e all'intero Piemonte. Anche la città di Torino, il sindaco della città, persone politiche che con Ugo hanno discusso e si sono confrontate sul piano delle idee, ne hanno riconosciuto il ruolo. Non a caso Ugo Martinat ha proseguito l'impegno anche nel Consiglio comunale di Torino, abbinandolo all'impegno politico parlamentare. È stato uomo della battaglia politica in anni difficilissimi. Ha iniziato il suo impegno politico in anni in cui collocarsi a destra era una scelta di coraggio e difficile in una città che ha conosciuto - come tante parti d'Italia - momenti difficili che fanno parte di una storia per fortuna oggi consegnata al passato. Ugo, poi, è stato un dirigente e un militante di partito nel senso più nobile del termine, nelle responsabilità che ha ricoperto, nella militanza giovanile e in quella di partito, come ricordavo prima, nelle assemblee comunali nella sua crescita e nel suo percorso nel Parlamento. È stato uomo molto legato alla vita del Parlamento, a lungo anche Questore alla Camera dei deputati e quindi legato anche alla quotidianità della vita parlamentare. È stato poi dirigente politico e quindi - come è stato ricordato - membro del Governo sia dal 2001 al 2006, in un'attività dedicata soprattutto alla politica del fare e dell'intraprendere e alla realizzazione di tanti progetti, che poi - fino alla sua scomparsa - al Ministero delle attività produttive. Ugo è stato legato a tanti di noi. Con Gianfranco Fini, con Ignazio La Russa, con Altero Matteoli, con Pinuccio Tatarella e con tutti noi ha condiviso questo impegnativo ed esaltante percorso che, da quelle esperienze che ormai appartengono ad una storia lontana, ha portato fino alla nascita del Popolo della Libertà. Fino al giorno prima, nonostante un male che inesorabilmente lo ha

seguire il suo calvario fino all'ultimo, egli ha discusso di cose politiche, del congresso che simultaneamente a questo dramma si era aperto, dell'organizzazione del nuovo partito, dimostrando fiducia in un destino (che forse sperava fosse più clemente), ma, soprattutto, consapevole che la sua esistenza di uomo pubblico di uomo dell'impegno politico era la sua vita, sostanzialmente e fino all'ultimo istante: dico ciò senza alcun retorica. È stato un uomo che ha condiviso ogni scelta e l'ha sempre condivisa con disciplina, quando era pienamente convinto e anche quando poteva nutrire qualche dubbio, ma seguendo il percorso di una comunità. Essendo uomo dell'azione e del fare, ha fondato radio, ha creato giornali e ha consentito a nuove generazioni di dirigenti politici di schierarsi, di crescere e di arrivare fino all'esperienza del Parlamento. Noi lo ricordiamo in questo modo: un uomo leale nella sua appartenenza a una comunità politica, un uomo che ha condiviso tutti i percorsi

questo lutto, ma a nome di tutto il Parlamento e di tutto il mondo politico, salutiamo con grande rimpianto (ma anche con la gioia di salutare un uomo che è stato un esempio) la scomparsa di Ugo Martinat, il cui ricordo certamente non si dissolverà.

e con lui aveva - se non condiviso le battaglie - condiviso il territorio, ai problemi del quale, ciascuno con le proprie idee e per la propria parte politica, cercavano con successo di dare risposte. Ugo era appunto una persona che dava risposte. sua caratteristica principale era innanzitutto l'affidabilità: a Ugo potevi affidare la tua vita, le tue idee, la tua amicizia, anche i tuoi soldi se per caso avessi avuto bisogno di affidarli a qualcuno, e potevi essere sicuro che lui avrebbe fatto esattamente quello che ti aveva detto e quello che ti aspettavi lui

un uomo tenace, riservato, un uomo che dà un grande valore all'amicizia ma che non ha bisogno di fronzoli per dimostrarla: sai che la

il responsabile, il presidente della Giovane Italia (qualcuno di voi sa che era l'organizzazione giovanile del Movimento Sociale) e poi del Fronte della Gioventù; siamo stati insieme coordinatori regionali giovanili, lui di Torino e io di Milano, poi presidenti provinciali del nostro partito di allora, il MSI, infine, i coordinatori regionali del Piemonte e della Lombardia di Alleanza Nazionale. Ugo era già diventato deputato, molto prima di me, e con lui ho condiviso una battaglia entusiasmante, che fu quella che portò Fini prima ad essere il segretario del Movimento sociale italiano e poi, insieme al nostro capo - chiamiamolo così

compiere una metamorfosi e diventare uomo delle istituzioni, uomo di governo, uomo delle responsabilità, uomo del fare e non solo uomo del contrastare. Ecco, Ugo ha svolto tutti questi ruoli con la stessa coerenza, con la stessa costanza, con la stessa

(la sua compagna d'amore di ora ci ha detto che sono stati gli unici dieci minuti del suo ultimo giorno di vita in cui non sembrava fosse ammalato), ha parlato con noi del presente, dell'oggi e del domani. Ha parlato con noi di chi secondo lui fosse più opportuno che facesse il coordinatore o il vice coordinatore di questa o di quella città della sua Regione.

che il percorso terreno che gli restava non fosse lunghissimo, ma con la mente era già proiettato al domani, a quando non ci sarebbe stato, perché sapeva che la vostra amicizia, il vostro ricordo e la nostra attività politica sarebbero stati una prosecuzione della sua vita. Così lo salutiamo. Grazie, Ugo, per quello che hai fatto per noi.

Grazie,

Signora Presidente, questa sera discutiamo di una questione straordinariamente importante, e lo vogliamo fare non per sancire un nostro punto di vista, né per cristallizzare una nostra posizione, ma per offrire un contributo, affinché il nostro Paese sappia partecipare allo sforzo che l'umanità deve compiere per risolvere la minaccia, che grava sull'umanità stessa, determinata dai cambiamenti climatici, la cui dimensione non può essere certo misurata con gli strumenti congiunturali che segnalano i decimali di incremento o di decremento delle

sono la conseguenza più diretta di fattori spinti di antropizzazione e di modificazione degli equilibri naturali quindi conseguenza del nostro modo di vivere e di produrre, del nostro modo di guardare al presente e al futuro. Oggi torna di grande attualità quella definizione di sviluppo sostenibile che vuole affidare alla responsabilità dell'oggi il compito di non impedire alle future generazioni di poter compiere le scelte che oggi stiamo compiendo noi e di disporre dei beni, delle opportunità, degli strumenti di conoscenza e delle materie di cui oggi disponiamo, perché le future generazioni possano fare altrettanto con quelle che seguiranno. La discussione sul clima oggi incrocia la discussione più generale sulla grave crisi produttiva e sulla recessione che investe tutte le economie mondiali: non è un caso che i grandi Paesi, proprio in queste ore, affrontando i problemi della ripresa economica e dello sviluppo, alludano anche a tali questioni; così come non è un caso che siano già stati previsti e definiti importanti appuntamenti internazionali, per discutere su come fronteggiare i cambiamenti climatici, con una platea di adesione e di partecipazione diventata più numerosa non solo per effetto delle decisioni del presidente Obama, ma anche che per la consapevolezza manifestata dai Paesi emergenti, che ritengono di assumere questo tema tra le proprie priorità e ritengono che anch'essi abbiano dei doveri da assumere rispetto a tale grave minaccia. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi si approderà alla definizione di una nuova agenda, di un nuovo impegno internazionale, per attualizzare gli impegni assunti a Kyoto e rispetto ai quali il nostro Paese segnala ritardi che hanno anche determinato una deroga rispetto agli impegni, assunti in sede comunitaria, circa il raggiungimento dell'obiettivo segnalato e conosciuto come "20-20-20". la deroga assentita all'Italia, e talvolta proposta come un grande successo, potrebbe rappresentare una grave minaccia per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese se essa venisse vissuta con un senso di irresponsabilità rispetto alla necessità del fare. E potrebbe rappresentare anche l'inconsapevolezza rispetto a questa straordinaria opportunità, che oggi i Paesi più accorti dell'Europa e del mondo e la nuova amministrazione americana intendono assumere per determinare una nuova fase dello sviluppo e della crescita economica, maggiormente caratterizzata dalla capacità di mettere a valore la conoscenza, i saperi e l'uso appropriato delle nuove tecnologie. La lotta al cambiamento climatico quindi, una potente occasione per la crescita e lo sviluppo economico, se noi sappiamo trasformare, appunto, questa criticità in una straordinaria opportunità. il nostro Paese ha già avviato, nel corso degli anni passati, un processo che è stato segnato anche da pronunciamenti unanimi proprio di questo ramo del Parlamento, quando alcuni anni fa, in relazione agli impegni relativi alla realizzazione degli obiettivi di Kyoto, fu approvato un documento unitario.

del benessere delle persone e, quindi, della garanzia della salubrità ambientale costituisce un motore eccezionale per il rilancio della nostra economia. Per questo è importante che il nostro Paese non giochi più in difesa; per questo è importante che il nostro Paese metta in campo quella straordinaria capacità che ha saputo in tante circostanze mettere in evidenza, per approdare a risultati importanti, utilizzando i saperi e il patrimonio di conoscenze e di capacità tecnologiche che la nostra industria è in grado di mettere in campo. In questa direzione, i progetti strategici di "Industria 2015", relativi all'energia sostenibile e alla mobilità sostenibile, rappresentano, come è evidente a tutti, una straordinaria opportunità di crescita e di sviluppo. Gli stessi orientamenti comunitari, non solo quelli relativi alla descrizione dei principi, ma anche quelli relativi alla allocazione delle risorse, vanno in questa direzione. Oltre un terzo del bilancio comunitario per i prossimi anni è destinato a sostenere processi di crescita e di sviluppo caratterizzati dalla sostenibilità ambientale. L'Unione europea impegna gli Stati membri ad utilizzare le risorse del bilancio per promuovere nuovi posti di lavoro verdi. Per questo noi non dobbiamo sciupare questa opportunità, allentando l'impegno o eludendo gli impegni; che la flessibilità accordataci possa accompagnare un processo in grado di recuperare il ritardo sin qui accumulato e di rimetterci nella condizione di guadagnare quel ruolo di prestigio e di punta che è possibile recuperare valorizzando il complesso dei patrimoni di conoscenze e di capacità operative di

che il Governo si impegni, con il supporto del Parlamento, in un'azione che sia fortemente caratterizzata da questa politica, perché riteniamo che questa politica serva alla preservazione degli equilibri naturali, ma anche a superare le situazioni di grave difficoltà nelle quali oggi ci troviamo ad operare.

Lo scopo di questa mozione sulla straordinariamente complessa e importante questione dei cambiamenti climatici è uno solo: chiedere al Governo di supportare e promuovere a Bruxelles un atteggiamento non dogmatico. Purtroppo, le recenti prese di posizione della Commissione europea sull'argomento, nella loro assoluta certezza dell'attribuzione della responsabilità del riscaldamento globale in atto soprattutto all'anidride carbonica antropogenica, non sono apparse affatto allineate a questo doveroso atteggiamento non dogmatico. La questione del clima è prima di tutto una questione scientifica. E la scienza, quella vera, è sempre non dogmatica, non ammette *ipse dixit*, è aperta agli approfondimenti, si ispira unicamente ad un totale amore per la verità. A scanso di equivoci, vorrei comunque fare una premessa. Noi del PdL siamo pienamente consapevoli del fatto che la terra è la nostra astronave, senza alcun possibile ricambio. La Terra va perciò tenuta pulita e passata alle future generazioni così ricca di vita e aperta alla vita come l'abbiamo ricevuta. Siamo perciò decisamente favorevoli ad una politica di sviluppo sostenibile e, in particolare in campo energetico, al risparmio energetico e allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Ma tutto questo con equilibrio, senza eccessi fondamentalistici, senza alcun catastrofismo. Due parole sull'estrema complessità del clima sul nostro pianeta. Oltre il 70 per cento della superficie terrestre (511 milioni di chilometri quadrati) è ricoperto dagli oceani, con potenti correnti oceaniche che veicolano verso i poli gigantesche quantità di calore. Il clima è sostanzialmente determinato dal Sole, sia mediante la possente radiazione elettromagnetica centrata nel visibile (circa 1.365 watt al metro quadrato), sia mediante un non trascurabile (ma spesso trascurato nelle valutazioni) vento solare formato da particelle elettricamente cariche. L'atmosfera gassosa che circonda il nostro pianeta è importante, come evidenziano il valore della pressione (1 chilogrammo per centimetro quadrato circa) e lo spessore (decine di chilometri), ed è animata da un complesso sistema di circolazione che veicola verso i poli enormi quantità di calore. Nella determinazione del clima hanno rilevanza il grande effetto stagionale, dovuto all'inclinazione di circa 23 gradi dell'asse di rotazione terrestre rispetto al piano dell'eclittica, dell'eclittica, le calotte polari fredde, in particolare l'Antartide, e il ciclo dell'acqua (con l'evaporazione dagli oceani, il trasporto mediante la circolazione atmosferica, la condensazione del vapore in sistemi nuvolosi, la precipitazione sotto forma di pioggia o neve). Nell'atmosfera gioca un ruolo cospicuo la presenza di anidride carbonica, la cui concentrazione è attualmente poco più di 380 parti per milione, cioè lo 0,38 per mille 0,38 per mille (mentre era di 280 parti per milione all'inizio dell'era industriale). Senza anidride carbonica la vita sul nostro pianeta non potrebbe esistere.

Questo effetto è in gran parte dovuto al vapor d'acqua, ma in modesta parte anche all'anidride carbonica (con molto minori contributi di altri gas). Da notare che il contributo dell'anidride carbonica è già in saturazione all'attuale concentrazione: un raddoppio di questa concentrazione produrrebbe un ulteriore effetto serra assai minore di quello finora prodotto dall'anidride carbonica stessa. Importanti aspetti della fisica e della chimica del clima non sono ancora sufficientemente conosciuti dalla scienza. Ad esempio, la formazione ed il ruolo il ruolo energetico delle nuvole, l'influenza del Sole e delle variazioni della sua emissione sul clima, in particolare del vento solare. Nella storia del nostro pianeta il clima è sempre variato per effetto delle più varie cause, non tutte conosciute. Ad esempio, la vicina Libia, attualmente drammaticamente carente d'acqua, anni fa, nell'epoca greco-romana, ne abbondava, come evidenziano i resti archeologici delle ricche terme di Leptis Magna e di Sabrata e delle terme private delle ville romane sulla costa. A Palmira, ora nel deserto siriano, fiorì oltre duemila anni fa una ricca civiltà sostenuta da una fiorente agricoltura. Migliaia d'anni fa l'intero deserto del Sahara era riccamente popolato di flora e fauna. La mozione raccomanda al Governo di intervenire con urgenza presso la Commissione europea e i Paesi del G8, del G8 + 5 e del anzitutto che una parte consistente e sempre più crescente di scienziati studiosi del clima non crede che la causa principale del peraltro modesto riscaldamento dell'atmosfera terrestre al suolo finora osservato (compreso fra 0,7 e 0,8 gradi centigradi) sia da attribuire prioritariamente ed esclusivamente all'anidride carbonica di emissione antropica. In sottolineare che le previsioni climatologiche a lungo termine, attualmente effettuabili mediante complicatissimi programmi di calcolo nei migliori centri di ricerca del mondo, sono ben lontane dall'essere affidabili, non essendo ancora sufficientemente conosciuti gli effetti climatici dovuti ad importanti elementi della fìsica terrestre, quali ad esempio nuvole, vulcani, oceani, particolato atmosferico, eccetera, nonché gli effetti climatici delle variazioni cosmiche e solari, e non essendo stati adeguatamente sperimentati e testati su affidabili serie storiche di dati climatologici gli estremamente complessi modelli di calcolo utilizzati per tali previsioni. altresì rimarcato come non sia ancora affatto chiarita la dipendenza della temperatura media dell'atmosfera terrestre al suolo dalla concentrazione dell'anidride carbonica nell'atmosfera. va osservato che, se pure vi fosse, a seguito dell'aumento della concentrazione dell'anidride carbonica nell'atmosfera, un aumento della temperatura terrestre al suolo, i conseguenti danni all'ambiente, all'economia e all'incolumità degli abitanti del pianeta sarebbero molto inferiori a quelli previsti nel rapporto Stern continuamente citato nei documenti della Commissione europea. suggerire come, piuttosto che avviare un costosissimo e probabilmente velleitario sforzo di mitigazione del riscaldamento globale in atto, più proficuo potrebbe essere destinare le risorse disponibili, inevitabilmente limitate, all'adattamento a tale riscaldamento e alla promozione di interventi sul territorio finalizzati all'efficienza energetica, all'edilizia ecovirtuosa, all'eliminazione dell'inquinamento ambientale da emissioni nocive e così via. va poi sottolineato che gli obiettivi intermedi e le relative sanzioni introdotte dal Protocollo di Kyoto e dal cosiddetto Accordo 20-20-20 tendono per loro natura a soffocare la dinamica degli investimenti in ricerca, sui quali si deve invece fare un grande sforzo epocale, poiché dalla ricerca possono venire soluzioni straordinariamente importanti per risolvere il problema del buon utilizzo delle risorse disponibili nel pianeta. In settimo luogo, occorre segnalare che il livello dell'acqua negli oceani non sta aumentando a ritmo preoccupante; che i ghiacciai basati su terraferma nelle calotte polari non si stanno sciogliendo; che il numero e l'intensità dei cicloni ed uragani tropicali non sta aumentando; che negli ultimi dieci anni la temperatura media al suolo dell'atmosfera terrestre non risulta aumentata; che secondo gli oceanografi non vi è alcun rischio di blocco della corrente del Golfo;

La mozione chiede, infine, che venga mantenuta la linea già espressa dal Governo in occasione della stipula della ripartizione degli oneri per il cosiddetto Accordo 20-20-20, in particolare per ottenere una attenuazione

Signora Presidente, mi rivolgo ai colleghi per cercare di dare una spiegazione a questa mozione che riguarda il clima. Quando parliamo di un argomento

Abbiamo cercato di non fare assolutamente questo. Abbiamo cercato di essere concreti in maniera tale che, se la mozione verrà approvata, si possa cercare di raggiungere qualcosa di concreto. La mozione è ispirata completamente e in maniera strutturale ad una piena sostenibilità ambientale e anche ad azioni concrete aventi la funzione di essere un punto di partenza, una base,

andate in contrasto. Dobbiamo puntare essenzialmente sullo sviluppo e sul potenziamento delle energie rinnovabili e sulla riduzione delle immissioni. Oggi notiamo con piacere e soprattutto con soddisfazione che la politica degli Stati Uniti sta adottando questa nuova filosofia che, sappiamo tutti, è vincente. Mi riferisco allo Mi riferisco allo sviluppo sostenibile e alle energie alternative; è una filosofia che sicuramente è, ma soprattutto sarà per il futuro un punto di partenza e un traino per le nuove economie. Questi sono temi vincenti per noi, per il futuro del nostro pianeta e per l'ambiente. Chiaramente quando parliamo di noi, di ambiente e del nostro futuro inevitabilmente il nostro pensiero va ai nostri figli.

abbiamo parlato semplicemente di energia rinnovabile, di sviluppo sostenibile e di modernizzazione ecologica per il rilancio dell'economia.

comprendere tutti i danni che sono stati fatti nel passato. La nostra storia, purtroppo, porta tanti esempi di sviluppo non sostenibile: basti pensare al grande sviluppo delle nostre zone industriali che, in maniera selvaggia, hanno devastato i nostri territori e ai grandi esempi di inquinamento, sia dei nostri mari

ha impostato la sua campagna elettorale e la sua azione di Governo sull'azione sostenibile e la modernizzazione ecologica dell'industria. Credo che anche noi, che da parecchio tempo parliamo di questo argomento, dobbiamo lavorare fortemente in questa direzione. Tutta la nostra industria ha una tecnologia che, purtroppo, è ancora molto legata al passato: abbiamo una redditività dei macchinari presenti nelle nostre industrie che non è al massimo per quanto riguarda i termini di rendimento. Su tale fronte, di lavoro ne possiamo fare sicuramente molto. Parlando di lavoro, per il rinnovamento del nostro parco macchine per quanto riguarda

argomento di grande attualità, soprattutto in questi ultimi mesi, relativamente alla modernizzazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento delle nostre abitazioni: anche questa è una grandissima opportunità, che dobbiamo cogliere, però, nella giusta versione della sostenibilità, nella visione di un miglioramento per quanto riguarda la coibentazione di queste abitazioni e strutture. Dobbiamo cogliere l'occasione

tutti dobbiamo attingere come esempio per quanto riguarda lo sviluppo futuro delle nostre abitazioni. Credo si sia capito che dobbiamo essere rispettosi dell'ambiente in cui viviamo e per far ciò basta seguire una regola molto semplice,

Credo che, attraverso questi presupposti, anche la nostra economia, che sta attraversando un momento sicuramente difficile, riceverà nuovi e sostanziosi stimoli, che ci permetteranno

Se imposteremo il futuro con questi nuovi concetti e criteri, credo che l'umanità futura, ma soprattutto i nostri figli, ci ringrazieranno.

Qui è in oggetto un argomento abbastanza stringente, ossia la differenza - crescente e preoccupante

L'insieme della comunità scientifica a livello mondiale, però, ha molti dubbi all'interno della ricerca, ed è giusto che sia così, ma ne ha pochi sul fatto che la tendenza ci esponga a pericoli di grosso rilievo. Quindi, c'è un punto di vista della comunità scientifica che perfeziona l'analisi e scopre nuovi elementi di precisazione di un pericolo globale: basta dare un'occhiata a qualsiasi sito, ma - meglio ancora - andare nelle biblioteche e confrontarsi con i centri di ricerca veri, per scoprire che ve ne dozzine e dozzine di specializzatissimi, che si interrogano su questi fenomeni e non hanno mai la pretesa di dire la verità, ma sempre semmai la tendenza ad accumulare fonti di dubbio e approfondimento.

dalla rivoluzione industriale in poi, è diventato prepotentemente un agente ecologico di straordinaria e forse inarrestabile potenza. E questo si traduce anche in influenza sui fenomeni climatici.

l'atteggiamento della maggioranza, la quale presenta una mozione che, dopo alcuni svolazzi, sostanzialmente tende a ridurre, quasi a vanificare,

di un rischio crescente in rapporto alla modificazione della struttura chimica dell'atmosfera, con elementi invasivi che produrranno un aumento preoccupante dell'effetto serra

tutte in ascesa

anche all'uso delle fonti energetiche fossili (combustione del petrolio, del carbone e così via). Di fronte a questo tipo di impulso è abbastanza curioso che un Governo - l'unico in Europa - adotti un atteggiamento di sottovalutazione sistematica.

la documentazione parla da sé: c'è un aumento del pericolo e c'è la necessità di fronteggiarlo, se non altro in base al criterio di precauzione. Si potrebbe anche avere il dubbio sistematico

cominciare a ricorrere sistematicamente a tutte le forme di energia rinnovabile; dovremmo inventare un tipo di produzione in rapporto all'incremento di questo tipo di necessità. c'è perfino una speranza di sviluppo economico, in senso stretto, all'interno della logica di precauzione. Mentre, da un lato, c'è la dissipazione finale delle risorse

cento dei consumi energetici del pianeta derivano da combustibili fossili (petrolio, gas e carbone) ed al loro consumo è collegato il problema relativo all'emissione di anidride carbonica, la cui concentrazione in atmosfera è considerata la causa principale dei cambiamenti climatici. Non intendo avventurarmi in una discussione su un tema certamente interessante, ma che implica la conoscenza tecnica e scientifica di fatti e dati che esulano dal compito e dal novero delle nostre conoscenze, ma il dato centrale è che, se un Paese come gli Stati Uniti e un presidente neoeletto come Obama orienta le politiche economiche anticrisi verso una ripresa cosiddetta ecosostenibile, una ragione ci deve

l'aiuto che il Presidente degli Stati Uniti ha concesso alla più grande casa automobilistica statunitense, la General Motors, è condizionato dall'accordo con la FIAT secondo cui si prevede

la promozione di un *fo**rum* sulla sicurezza energetica e contro i cambiamenti climatici che si terrà nel corso del G8 di luglio in Italia.

il nostro Governo, l'Unione europea debbano mettere in campo per affrontare al meglio la crisi e non vi è dubbio che di queste politiche e di questo pacchetto deve far parte anche la scelta chiara e netta su alcune questioni che attengono alle politiche energetiche del nostro Paese, da troppo tempo dimenticate e affrontate timidamente, sicché non siamo messi nelle condizioni

fanno crescere i nostri costi di produzione. Quindi, in buona sostanza, l'assenza di una strategia e di una politica decise, che portino a scelte precise e a tutto campo, rischia di penalizzarci due volte: non ci fa né, da un lato, protettori dell'ambiente, né, dall'altro, investitori sui temi energetici, aspetto che invece è diventato una priorità per le evidenti ragioni che

È un convitato di pietra perché su questo tema, al di là di un accordo e di un'intesa dai contenuti vaghi del nostro Paese con la Francia Francia e di una serie lodevole di petizioni di principio e di qualche norma agevolativa delle procedure proposte ed approvate da questo Governo, si è ancora in una fase iniziale rispetto all'esigenza di una svolta nel settore della ricerca e dello sviluppo del nucleare che, per essere chiari, rappresenta per l'Italia la più grande occasione per affrancarsi nel fabbisogno energetico da Paesi terzi e rappresenta, nel medio e nel lungo periodo, la soluzione ai tanti problemi che oggi ricadono sulle famiglie italiane con riferimento al costo delle bollette energetiche e quant'altro. La prova provata di ciò nasce dalla circostanza che Paesi come il Kuwait e come la Svezia hanno aperto al nucleare e dalla circostanza che il presidente Obama, che viene oggi citato solo perché considerato esclusivamente un ecologista, ha stanziato 18 miliardi e mezzo di dollari per il nucleare. C'è una presa di coscienza forte da parte di tantissimi Paesi, anche di Paesi produttori di petrolio come il Kuwait cui accennavo prima, che ci dovrebbe far riflettere ed anche accelerare una inversione di tendenza nel nostro Paese su questo tema. tema che va coniugato con quello relativo allo sfruttamento delle energie da fonte rinnovabile; un tema che è collegato anche all'incentivo nel settore dell'edilizia. Chi vi parla nel nostro Gruppo non si è mostrato contrario alle proposte del Governo sul piano sul piano casa e sulla necessità che il nostro Paese sia messo nelle condizioni di poter ammodernare il proprio patrimonio immobiliare rendendolo compatibile con le nuove previsioni e con i nuovi sistemi che determinano un risparmio energetico, posto che ad esempio vi sono stime che ci indicano che il settore edilizio è responsabile di circa il 40 per cento dei rifiuti prodotti nei Paesi europei e di un elevato inquinamento. Credo che questo tema, come quello del sequestro dell'anidride carbonica che è affrontato diffusamente nella nostra mozione, così come il tema relativo allo stoccaggio dell'energia, agli incentivi

realizzazione degli impianti di produzione di energia eolica sono un complesso di disposizioni e di interventi che devono essere oggetto di una scelta chiara e di una politica complessiva del Governo

che credo sia comune un po' a tutti, che dovremmo anche assumerci la responsabilità di dire che un Paese consapevole non può fare scelte di politica energetiche, anche pesanti, anche importanti, molto responsabili, attraverso La nostra Carta costituzionale in questo senso va corretta: non è possibile che vi sia una scelta strategica nazionale verso il nucleare, fatta ad esempio da un Governo, quando poi le singole Regioni, chiamate a collaborare in una strategia che è nazionale, perché riguarda la produzione di energia che è che è un interesse esclusivamente nazionale e non regionale, si oppongono stabilendo che in quel territorio non si possa fare una centrale nucleare, come se fosse un problema legato solo ed esclusivamente a quella porzione di territorio e non invece agli interessi strategici del Paese. Signora Presidente, dobbiamo avere il coraggio

La crisi che noi viviamo accelera scelte chiare e nette in questo settore. In tal senso va la nostra mozione e ci auguriamo che se ne colga lo spirito costruttivo e propositivo.

ormai da tempo l'*iter* del cosiddetto pacchetto clima-energia e ho rappresentato il Senato italiano presso la Commissione europea nel novembre scorso a Strasburgo. Ritengo che l'equilibrata posizione assunta dall'Italia nelle varie fasi della discussione del pacchetto 20-20-20, tra l'altro apprezzata e a volte seguita da altri Paesi membri, continui a manifestarsi sia nello studio che nell'impegno. Voglio ribadire che la nostra politica attuale deve tendere al rispetto degli accordi presi, seppur in considerazione di una elasticità che permetta a noi e agli altri Stati una sostenibilità delle misure ed un accettabile rapporto tra i costi attuali e i benefici futuri. Questo significa che dobbiamo avere ben presente la situazione climatica, le percentuali dei gas serra, la valutazione delle fonti di energia e del loro impatto ambientale. Non abbiamo mai sottovalutato l'impatto climatico dello sfruttamento energetico qual è stato sinora, ma neanche, secondo me, dobbiamo dare cieco credito a studi catastrofisti, peraltro ormai piuttosto datati. Tra il 1990 e il 2005 l'Europa ha dato un significativo contributo alla riduzione di emissioni di CO2 perché i Paesi membri, a fronte di una crescita del PIL del 2,1 hanno comunque assicurato una riduzione delle loro emissioni di circa il 3 per cento, mentre nello stesso periodo le emissioni di CO2 sono aumentate del 20 per cento negli USA e quasi raddoppiate in Cina. Senza dubbio il Governo italiano si muove nell'interesse della salvaguardia della popolazione, del territorio e del clima, sia rivolgendosi direttamente agli italiani nella loro funzione di guidatori di auto (come ha fatto di recente il ministro Scajola), dando consigli pratici per risparmiare carburante e ridurre le emissioni di gas da parte delle autovetture, sia stipulando l'accordo fatto dal presidente Berlusconi con il presidente Sarkozy sul nucleare, che tanti esperti hanno ormai riconosciuto come la migliore fonte di energia pulita disponibile. Voglio ribadire il fatto che noi europei possiamo fare tutto il possibile, e anche di più, per la salvaguardia del pianeta, ma se altri grandi Paesi si muovono su strade diametralmente opposte si rischia di vanificare tutti gli sforzi ed i sacrifici. Dallo stesso Congresso USA arrivano reazioni molto tiepide alle proposte del presidente Obama e, a quel che ci risulta, la sua amministrazione pensa ad un obiettivo molto più modesto rispetto a quello che si prefigge l'Unione europea. È significativo il fatto che il presidente Obama, nell'invitare i *leader* di 16 grandi potenze a Washington per la creazione di un *Forum* su clima e energia, abbia scritto al presidente Berlusconi per organizzare un vertice in Italia, che si terrà a luglio alla Maddalena in concomitanza con il G8, e per avere il suo aiuto per riattivare il *Major Economies* *Forum* sull'energia e i cambiamenti climatici. Per questo, ben venga un nuovo monitoraggio, basato su più nuove e sofisticate tecnologie, che ci dia un quadro più puntuale e aggiornato del precedente e che ci faccia prendere decisioni di peso senza sottoporre i cittadini a sacrifici pesanti quanto spesso inutili.

un dibattito che ha avuto anche un esito propositivo, tanto da confluire addirittura su una mozione congiunta tra maggioranza e opposizione. È normale, verrebbe da dire, perché sono temi per i quali il dibattito si svolge non soltanto dentro queste mura e quindi, per fortuna, anche le soluzioni non possono che essere globali, transnazionali e anche trasversali rispetto ai Gruppi parlamentari. Il Senato però oggi ha deciso di trasformare il dibattito sul clima, sul riscaldamento globale e sulle possibili azioni del Governo su queste tematiche in qualcosa di surreale, se non ridicolo, a causa della mozione del Popolo della Libertà, vista e rivista - tra l'altro - fino alla terza versione da poco consegnataci. Affrontare temi di questa portata, anche con approcci critici rispetto a quelli tradizionalmente inquadrabili come ambientalisti, non può però scadere nella *pochade*. Abbiamo una mozione che bolla come Cassandre pericolose e catastrofiste una parte del mondo scientifico; insinua il dubbio - per poi negarlo - sul rapporto tra il riscaldamento globale e l'emissione di anidride carbonica da parte dell'uomo; ridicolizza la comunità scientifica e politica internazionale e poi, nella prima e seconda versione, annuncia perfino, in maniera ottimistica, che seppure esistesse seppure esistesse il riscaldamento globale, se ne ricaverebbero più benefici che altro. La terza versione lascia solo il dubbio, scompaiono però i benefici. Credo che, se da un lato la mozione della maggioranza si propone, dopo aver negato la realtà, di adattarsi

miliardi di persone nel 2050, una vera bomba demografica) siano spunto e occasione per lanciare una sfida per la crescita del Paese, per l'innovazione, per la competitività, per la modernizzazione. E il il nostro Governo, che si è contraddistinto per una battaglia di retroguardia, di rinvio, al ribasso in sede di Unione europea, invece che diventare protagonista su un punto importante quale potrebbe essere quello dell'efficienza energetica, ci propone queste soluzioni davvero di retroguardia.

Vi propongo una distinzione classica, che non è assolutamente inventata da me, tra i ritmi dei mutamenti naturali e i ritmi dei mutamenti di origine umana.

I cicli dei grandi mutamenti naturali sono quelli rappresentati dalle glaciazioni. Può essere interessante sapere che, nell'ultima glaciazione, il cui acme è datato intorno a 30.000-25.000 anni fa, quindi un tempo geologico relativamente molto recente, la diversità della temperatura media dell'atmosfera era tale che il livello del mare era 120 metri inferiore a quello attuale. Quindi, per esempio, dalla Toscana si poteva andare a piedi all'Isola d'Elba e questo spiega come gli aborigeni australiani siano arrivati in Australia: hanno varcato lo stretto di Torres, dove oggi c'è un mare bassissimo, senza navigare, perché appunto il mare era più basso della terra. è fissato l'inizio, scelto per convenzione, di un grande periodo di raffreddamento, che in soli 20.000 anni, quindi in un tempo geologico brevissimo, si rovescia in un processo di riscaldamento.

Questo tipo di processo è testimoniato da infinite prove, su cui non insisto, che però possono anche essere bellissime da osservare: penso alle morene glaciali, alle testimonianze paleontologiche e, soprattutto, a quelle paleoclimatiche, che sono spietate quanto a precisione. L'uomo, fino a quel punto, non ha avuto nessun ruolo se non quello di subire, come tutti gli altri esseri viventi, l'effetto delle alterazioni climatiche. Intorno a 5.000 anni fa, nell'*optimum* climatico, per generale ammissione storica, l'uomo ha cominciato a diventare un agente ecologico potente, tramite l'agricoltura, l'allevamento e il pascolo. Può sembrare un fenomeno di scarso peso, ma l'agricoltura mette allo scoperto i suoli, rovesciandoli; l'allevamento ne consuma il manto erboso; aumenta enormemente l'erosione,

fa. Questo tipo di ritmo può essere visto in modo più ravvicinato: vi propongo dunque di considerare un ritmo più stringente nell'età storica. Gli storici del paleoclima hanno accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, che c'è stato caldo nella età romana, freddo durante la crisi del mondo antico,

locale. Questo è il ragionamento che dobbiamo fare. Abbiamo di fronte una testimonianza materiale di incremento progressivo del riscaldamento terrestre di fronte a questo, noi dobbiamo ragionare in termini pragmatici. La soluzione pragmatica è molto semplice: rinunciare alla moltiplicazione, peraltro solo finale (perché oramai siamo agli atti finali), del consumo dei combustibili fossili; prendere decisamente la linea della costruzione di tutte le fonti alternative di energia;

La situazione è molto semplice: noi siamo gli attori, in gran parte largamente involontari (l'edonismo privato è infatti un soggetto involontario),

Quindi, l'uranio è raro. Inoltre, l'uranio di cui disponiamo oggi non rappresenta una soluzione energetica convincente. Le quattro centrali nucleari che Berlusconi vuol farci comprare dalla Francia sono una patacca; sono centrali nucleari vecchie, non insegnano nuova tecnologia a nessuno, non danno sicurezza sotto il profilo (che noi vorremmo garantire) di tipo progressivo per il futuro, sono tutt'altro che nucleare di quarta generazione e non sono nemmeno un'introduzione all'appropriazione da parte nostra del nucleare di quarta generazione. Sono un prodotto vecchio, laterale e marginalizzato, che noi compreremo e di cui, probabilmente, si avvarrà soltanto l'Enel, che potrà lucrare sull'operazione sotto il profilo puramente contabile. Per il resto, il guadagno del nucleare è assolutamente discutibile

trovare una vera soluzione al problema delle scorie delle lavorazioni nucleari. Questo è un problema che una comunità consapevole dovrebbe porsi, senza avere la fissazione di pensare

In Italia non esistono spazi vuoti praticabili. Esiste una struttura montagnosa che occupa più della metà dello spazio, la popolazione è diffusa in modo più sparso le coste, che rappresentano l'unico posto dove si potrebbe captare l'acqua, sono abitatissime e sono, a loro volta, una fonte straordinaria di un'economia di altra natura.

questo dibattito rischia di diventare un serio infortunio politico, in vista soprattutto delle responsabilità internazionali che l'Italia è chiamata ad assolvere e soprattutto della guida del G8, che si concluderà con il vertice nell'isola nell'isola della Maddalena, oltre che con un vertice sui temi ambientali e con uno sui temi energetici. Quindi, farò un intervento solo di merito politico, partendo dalla premessa che è del tutto legittimo che ci siano in quest'Aula opinioni, desunte dal dibattito scientifico, anche divergenti, certamente articolate e diverse, ma non è possibile che il Parlamento della Repubblica italiana, nella sede dell'Assemblea del Senato, prenda una posizione politica impegnativa contrastante con quella di tutti i grandi Paesi del mondo, da qualunque Governo siano retti quanto a segno politico. E a questo brevemente mi dedicherò. La posizione sostenuta dal senatore Possa poco fa, che è agli atti del Senato, e le tre diverse successive versioni forse ne arriverà una quarta - della mozione predisposta dalla maggioranza non è adesso nostro compito discuterle dal punto di vista scientifico. C'è un aggiornamento costante, senatore Possa, che va in una direzione opposta a quella, pur rispettabile, da lei espressa. Cito soltanto la notizia che è stata diffusa tre giorni fa dalla stampa statunitense per cui il MIT, l'Istituto di tecnologia di Boston, ha aggiornato nelle ultime settimane le sue proiezioni nell'ambito del modello di sistema globale integrato sul cambiamento climatico, che analizza e proietta i dati dal 1861 al 2100, con delle previsioni nettamente più più preoccupate e più critiche alla luce di una serie di fattori che, ripeto, evoco, ma non richiamo: risulta che un fattore di interazione moltiplicativa che riguarda i ghiacci, che riguarda il riscaldamento dei mari, che riguarda una serie di fattori propri dell'atmosfera sta portando a previsioni peggiori, più critiche, più negative di quelle che sono alla base del quarto rapporto

politico, perché oggi il dibattito internazionale dà per acquisita la preoccupazione di natura scientifica e si sta orientando sulle risposte economiche, cioè su come la componente ambientale può diventare una risposta alla crisi E questo è il dibattito che avviene oggi molto più tra i soggetti economici e finanziari che in sede scientifica, ripeto, poiché si dà per acquisita una valutazione, nella quale convive naturalmente il dubbio, è presente un vivo dibattito, c'è un'attenta polemica, ma c'è anche una schiacciante determinazione dei soggetti scientifici. Come può il Governo italiano immaginare di guidare il G8 su una posizione come quella contenuta nella mozione che

assunta due anni prima dal precedente Governo conservatore ed ha proposto alla nuova amministrazione americana Obama un accordo per affrontare congiuntamente, con delle politiche incisive per ridurlo in modo spettacolare, l'inquinamento che contribuisce

il quale, nel suo discorso di insediamento ha assunto fortissime posizioni riguardanti il cambiamento climatico. Egli ha infatti dichiarato due mesi fa, al momento del suo insediamento, al problema del riscaldamento globale, di affrontare insieme la sfida ambientale e quella economica, assumendo una nuova *leadership* del nuovo Governo di impronta moderata e conservatrice giapponese. Il presidente

"C'è un'evidenza scientifica sostanziale fortissima che il cambiamento climatico cui stiamo assistendo è provocato provocato dall'uomo". Non è la dichiarazione di un esponente scientifico, ma di un esponente politico del maggiore Paese europeo nostro alleato, che siederà accanto a Berlusconi tra poche settimane nel vertice della Maddalena.

"L'evidenza scientifica è schiacciante. Anche se gli scienziati avessero torto non perderemmo nulla. È una responsabilità che ci dobbiamo assumere". l'Inghilterra, si conosce la posizione del Governo Brown, quindi quella che il primo ministro Brown porterà al vertice presieduto dall'Italia. Ma l'opposizione conservatrice sta sfidando Brown su una posizione ancora più impegnativa ed il *leader* dei Conservatori Cameron ha dichiarato (addirittura riprendendo una posizione, che ha definito visionaria ed anticipatrice, della signora Thatcher, nel suo ultimo discorso politico) che questo deve diventare uno dei punti qualificanti della politica di un eventuale Governo conservatore che subentrasse nel Regno Unito a quello

dai conservatori di Sarkozy. Vi leggo quanto il presidente Sarkozy ha detto in uno dei più importanti discorsi che ha fatto su questo tema: "La sicurezza del mondo è profondamente minacciata dai cambiamenti climatici. Oggi nessuno può più dire che non sapeva. Noi sappiamo." - dice Sarkozy - "Il punto centrale della politica ambiziosa che ci dobbiamo dare è la drastica diminuzione delle emissioni di gas serra. Questo punto non può più fare oggetto di dibattito.

serio) ad una lettera ricevuta dal presidente degli Stati Uniti Obama, l'altro convitato del G8, con cui gli aveva chiesto di tenere un vertice internazionale sui cambiamenti climatici alla Maddalena,

con gioia la richiesta di Obama di voler porre il tema dei cambiamenti climatici al centro del vertice della Maddalena. Oggi, il commissario europeo Dimas,

non è una buona cosa, né per l'economia, né per la sicurezza energetica, né per l'occupazione. Gli obiettivi europei" - dice - "sono sicuri e addirittura li dobbiamo rafforzare". Infine, Presidente, il ministro degli affari esteri Frattini - che rappresenta

e anche uno strumento di rilancio dell'economia. Questo dice oggi il Ministro degli esteri del Governo italiano. Vi pare possibile che il Parlamento italiano possa approvare una mozione che va esattamente nella direzione opposta agli impegni che l'Italia ha preso e difenderà in seno al G8, alla promessa che oggi ha fatto il Presidente del Consiglio al Presidente degli Stati Uniti invitandola a parlare su questi argomenti nel *summit* del G8 in Italia, alla Maddalena, e che il Ministro degli esteri oggi ha assunto come un tema di interesse comune e prioritario? Il mio invito non polemico e la mia conclusione sono che su queste materie dobbiamo cercare di trovare una convergenza nell'interesse del Paese.

in quella mozione, l'espressione politica. Ecco perché è il caso che ci si unisca, come è avvenuto a Montecitorio, signor Presidente, dove maggioranza e opposizione hanno votato uno strumento parlamentare per incidere sulla crisi economica con misure ambientali. Noi salutiamo anche l'intesa che c'è tra le Regioni e il Governo sul piano casa perché può essere una strada importante anticiclica per lo sviluppo economico, senza distruggere l'ambiente, e per creare una nuova generazione di edilizia biosostenibile. Reclamiamo dall'opposizione un piano di stimolo per l'economia che includa molto più fortemente le misure sostenibili dal punto di vista ambientale. Tutti questi argomenti, di fronte alla crisi economica, dovrebbero rappresentare motivo di impegno comune e di convergenza per cui l'opposizione dà la sua disponibilità al Governo. Non trasformiamo però il dibattito di oggi in un tardivo tentativo di riportare dentro una deliberazione del Parlamento - sarebbe legittimo se fosse un dibattito in un convegno - una linea che contraddice gli indirizzi della comunità politica internazionale che scaturiscono dalla larga convergenza della comunità scientifica. Per questo noi sosteniamo le diverse mozioni che portano avanti questa linea e invitiamo la maggioranza a un ripensamento radicale di quel documento che, invece, la contraddice, in questo sbagliando. Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, con la nostra mozione non abbiamo detto che il re è nudo: ci siamo limitati a dire

attribuendogli quanto è stato scritto per iniziativa parlamentare. E mi stupisco di vedere questa incapacità di riconoscere l'autentica origine parlamentare di questo documento proprio da parte di coloro che, quando il Governo adopera gli strumenti che la Costituzione peraltro prevede per arrivare alla rapida approvazione di provvedimenti, si scandalizzano per la presunta lesione dei diritti del Parlamento, che invece oggi sta agendo nella sede propria, con la piena consapevolezza di quanto sta facendo. Voglio aggiungere un altro elemento: la nostra mozione non è assolutamente in contrasto, anzi, sostiene le incontrovertibili esigenze di migliorare la sicurezza energetica del nostro Paese e dell'Europa, di aumentare l'efficienza energetica, di limitare gli sprechi e anche di andare verso una differenziazione delle fonti energetiche sia come tipologia delle stesse sia come luogo di provenienza, per il bene del nostro Paese e del nostro sviluppo. Tuttavia, abbiamo sentito il dovere di ricordare alcuni fatti incontestabili: quando si parla di consenso scientifico sul riscaldamento globale causato dall'uomo, si sta dicendo una cosa semplicemente falsa. Il *leader* della minoranza repubblicana nella Commissione ambiente e lavori pubblici del Senato degli Stati Uniti, negli scorsi mesi, un rapporto contenente le opinioni partitamente espresse da 650 scienziati di tutto il mondo, che non credono al riscaldamento climatico causato dalle emissioni delle dalle emissioni delle attività umane. A questi 650, nei soli due mesi seguiti a tale presentazione, se ne sono già aggiunti altri 60. Vorrei citarvi alcune di queste affermazioni, che - lo ripeto - sono oltre 700. «Le paure sul riscaldamento sono il peggiore scandalo scientifico della storia. Quando la gente verrà a sapere qual è la verità, si sentirà ingannata dalla scienza e dagli scienziati»: Kiminori Itoh, scienziato giapponese, membro dell'*International panel of climate change* (il famoso IPCC), che ha vinto anche parecchi premi scientifici internazionali. «Fino ad ora», dice Jarl Ahlbeck, un ingegnere chimico dell'università finlandese Abo Akademi, «le vere misurazioni non danno alcuno spazio a preoccupazioni su un futuro catastrofico riscaldamento del pianeta». Il fisico solare Pal Brekke, consigliere del Centro spaziale norvegese, autore di moltissimi articoli su questo argomento, ha detto che: «Chiunque afferma che il dibattito è chiuso e che le conclusioni sono certe ha

che fa sembrare gli scienziati scettici su questa teoria semplicemente una frangia trascurabile». E così via, ma ne aggiungo ancora tre:

E ancora, Takeda Kunihiko, vice cancelliere dell'Istituto di scienza e tecnologia dell'università Chubu, in Giappone, ha detto che: «Le emissioni di anidride carbonica non fanno alcuna differenza in un modo o nell'altro sul clima. Ogni scienziato lo sa, ma non è remunerativo dirlo». Un altro scienziato lo mette in luce in modo ancora più chiaro: del paleontologo Eduardo Tonni, dell'Istituto di ricerca scientifica di Buenos Aires, secondo cui: «Coloro che diffondono paure sul riscaldamento globale trovano la loro giustificazione nel fatto che queste paure generano l'erogazione di fondi».

sono state inopinatamente abbassate in modo da farle risultare più basse di quelle attuali. C'é poi un'altra tabella interessante che mostra l'andamento della temperatura negli ultimi dieci anni dalla quale emerge chiaramente che l'anno più

affermando che in un momento in cui si parla di 20 milioni di disoccupati in più nell'Unione europea, dove ancora nel mondo fame, malattie, violazione dei diritti umani affliggono centinaia di milioni di persone, pensare di investire centinaia di miliardi di euro finanziando attività la cui utilità è quantomeno dubbia, non è cosa opportuna. Chiediamo, prima di fare ulteriori passi, accertare quale sia la verità scientifica, non ascoltando soltanto i 52 scienziati dell'IPCC, ma anche le centinaia e centinaia di scienziati che hanno opinioni assai diverse.

devo riprendere ciò che ha detto nella sua introduzione il senatore Rutelli: evidentemente sono qui solo perché è il primo di aprile. Francamente, ritengo che la materia, per l'importanza degli argomenti che oggi debbono

Ciò premesso, è ovvio che non posso far altro che limitarmi a formulare una serie di considerazioni derivanti dall'esperienza pratica

dove notiamo cambiamenti nella fauna ed anche nella flora sottomarina derivanti da un innalzamento delle temperature dell'acqua. Più volte abbiamo che i fenomeni di precipitazioni violentissime estremamente localizzate, verificatisi nel corso degli ultimi anni nel nostro Paese, sono derivati sicuramente

un aumento di fenomeni negativi dal punto di vista meteorologico, sia in eccesso che in diminuzione delle temperature, che non hanno più i tempi di ritorno decennali o più che decennali,

naturali; infatti, è ancora troppo presto per poter emettere giudizi definitivi su questo genere di argomenti. È anche vero

che invece - come noto - è stata estremamente controversa ed ostacolata prima di essere definitivamente risolta. Per quanto riguarda il G8 che si terrà

riportare sul logo ufficiale del G8 una specie in via di estinzione, quale la tartaruga marina "Caretta Caretta", non è stato un mero esercizio teorico finalizzato solamente ad avere un riscontro

è impegnato su una politica di stretta osservanza delle buone regole ambientaliste: i "grandi della terra" useranno solamente energia

degli importantissimi ragionamenti e delle determinazioni che dovrete assumere, ma è qualcosa di concreto che il Governo sta portando avanti per mostrare

che Obama ha usato una penna prodotta dal mais per firmare l'accordo su carta riciclata, portando una maglietta prodotta dalla canapa e usando un microfono che utilizza energia elettrica fornita dal sole o dal vento

apprezziamo lo sforzo introdotto in questo dibattito su una visione diversa, sotto il profilo scientifico, dei temi che riguardano le emissioni e il riscaldamento della terra,

pericoloso introdurre temi di questa natura in un dibattito che invece ci porta a dover affrontare la questione energetica nel quadro delle politiche anticrisi e quindi anche con riferimento a ciò che

Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, mi pare che questo dibattito importante nasca come mera strumentalità e supporto per i prossimi impegni che

dovrò necessariamente entrare sul punto di quella presentata dai colleghi di maggioranza e che il senatore Malan ha detto essere una mozione parlamentare; io aggiungo che è una mozione parlamentare di ispirazione governativa, tant'è che è talmente cambiata che parte con un impegno e finisce in una mera raccomandazione; in pratica, svilendo il contenuto e il senso di una mozione parlamentare.

di andare contro la legge 1° giugno 2002, n. 120, votata dal Parlamento della Repubblica italiana che quel Protocollo ha ratificato. Quindi, chiede di violare i contenuti di una legge dello Stato, perché mostra di considerare i mutamenti climatici come una sorta di invenzione degli ambientalisti e di qualche scienziato, senza tenere presente che lo sforzo richiesto all'Italia nell'ambito del pacchetto clima-energia dell'Unione europea è sicuramente impegnativo e complesso, ma non può essere disatteso. Piuttosto che chiedere al Governo di formulare in sede europea solitarie richieste di rinegoziazione del *target* del pacchetto, l'Italia dovrebbe preoccuparsi maggiormente di tutelare le esigenze e gli interessi dell'industria italiana, senza rischiare un suo potenziale isolamento a livello internazionale. Se la posizione è quella espressa dalla mozione presentata dal senatore D'Alì e da altri senatori, è così. Noi riteniamo che il Presidente della Commissione ambiente, che è il primo firmatario di una mozione che dovrebbe rappresentare un po' il senso di quanto emerge nella stessa Commissione, avrebbe dovuto mantenersi

carica, piena, emblematica dell'ecoscetticismo che vi è nella maggioranza e nel Governo. Pensiamo pertanto di non poterla votare, mentre

ma non ci convince il richiamo al nucleare, in quanto siamo fermamente convinti che questa sia una follia come scelta, che peraltro il Parlamento ancora non ha fatto nonostante sia stato già siglato dal Presidente del Consiglio un patto bilaterale con il Governo francese. ai presentatori della mozione D'Alì e al Governo di cercare di trovare una sintesi virtuosa tra le diverse mozioni, che hanno tutte a cuore ‑ questo forse sì ‑ il bene ambiente, che in Italia viene spesso ferito da una serie di difficoltà, di mancate precauzioni

La mozione D'Alì, anche in modo provocatorio, mette in discussione una serie di questioni che hanno portato gli Stati ad aderire prima al Protocollo di Kyoto e, successivamente, ai negoziati per i vincoli dell'Accordo 20-20-20 e del *post* Kyoto. Tutti questi Protocolli e negoziati scaturiscono da relazioni di illustri scienziati che da anni studiano la climatologia e gli effetti delle emissioni. Ovviamente, la ricerca è in continua evoluzione e gli scienziati hanno in continua osservazione gli effetti climatici dovuti agli elementi della fisica terrestre, come le nuvole, i vulcani, le variazioni solari. Dal momento che una parte di questi scienziati e studiosi del clima si dimostrano scettici nei confronti della teoria dell'attribuzione del riscaldamento globale in atto alle attività umane e all'anidride carbonica di emissione antropica, tutta l'Europa deve tenere conto di ciò, ai fini della determinazione della propria politica ambientale ed energetica. Lo Stato ha il dovere di promuovere tutte le azioni possibili per un dibattito in materia, diretto ad approfondire la teoria sul riscaldamento globale. Sono infatti noti gli sforzi che devono compiere gli Stati membri, e in particolare l'Italia, per ottemperare al cosiddetto Accordo del 20-20-20, specialmente nell'attuale momento di crisi economica e finanziaria che si è abbattuta sul sistema globale e che richiede un'assunzione di responsabilità circa le politiche da mettere in atto per difendere e rilanciare l'economia dei Paesi. Peraltro, un'eccessiva attenzione agli effetti e mitigazioni del riscaldamento globale e alla riduzione dell'anidride carbonica rischia di far trascurare la promozione di interventi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento da inquinanti atmosferici come gli ossidi di azoto o le polveri sottili, che sono dannosissimi per la salute della popolazione e con effetti pesantissimi su territori con particolari caratteristiche geomorfologiche, come la Pianura padana. Per quanto concerne le mozioni Della Seta e Belisario, desidero far notare che il nostro Gruppo ha sempre dichiarato e proposto, con emendamenti presentati in varie occasioni, alcuni concetti base presenti negli impegni delle mozioni, tanto è vero che una serie di questi impegni fanno parte della mozione presentata dal nostro Gruppo. Mi riferisco, soprattutto, alla promozione dei legittimi interessi nazionali nel negoziato in sede europea sulle misure di lotta ai mutamenti climatici; al sostegno della ricerca, dell'innovazione tecnologica e del risparmio energetico; alla necessità di perseguire politiche innovative nel settore dei trasporti e della mobilità (anche per abbattere l'inquinamento da polveri sottili particolarmente i nostri territori); alle incentivazioni per la sostenibilità energetico-ambientale dei programmi edilizi. Si tratta di temi da sempre perseguiti dalla Lega Nord e dallo stesso Governo con le misure anticrisi. Chiaramente, però, non possiamo accettare i segni del catastrofismo profuso sull'intera mozione mossi dall'eccessiva persecuzione dello spettro del riscaldamento globale o votare impegni come quello di porre l'Europa all'avanguardia nel fronteggiare mutamenti climatici o di imporre vincoli aprioristici per la difesa dell'Accordo 20‑20‑20. Sono impegni che inevitabilmente finirebbero per penalizzare le nostre imprese, specialmente in questo momento di drastico deterioramento degli scenari macroeconomici internazionali, laddove lo Stato ha l'obbligo di trovare un punto di equilibrio conciliando l'esigenza di promuovere i sistemi produttivi, ovviamente in termini compatibili con la tutela dell'ambiente, ma anche con la strategia di non imporre agli stessi sistemi produttivi oneri eccessivamente gravosi. D'altra parte, non si può non tener conto di tutta la serie di vantaggi che può portare alla politica energetica del Paese un ritorno allo sviluppo dell'energia nucleare, anche per evitare che il nostro Paese resti fuori dai piani europei in materia.

per mitigarli - che in tutto il mondo vede impegnati destra e sinistra, maggioranze e opposizioni, Governi e comunità scientifica. Nel mondo c'è consenso scientifico sulla realtà dei mutamenti climatici e sulla loro parziale ma rilevante origine antropica. C'è concordia tra chi si occupa di questi temi anche sul fatto che i mutamenti climatici già in atto, e ancora di più quelli che arriveranno, se prevarrà l'immobilismo, rappresentino un danno gravissimo in termini sociali ed economici. nel mondo oggi c'è un crescente consenso politico - lo ha richiamato nel suo intervento il senatore Francesco Rutelli e lo ha anche documentato, riassumendo brevemente dichiarazioni e impegni di molti leader mondiali - sulla necessità di adottare strategie realistiche ma incisive per fronteggiare questo problema e sull'utilità di percorrere questa strada anche rispetto all'esigenza di rispondere alla crisi finanziaria ed economica di questi mesi. Le politiche per accrescere l'efficienza e il risparmio negli usi energetici le politiche per promuovere lo sviluppo delle energie pulite possono dare infatti al tempo stesso risposte decisive rispetto agli obiettivi di riduzione dell'impatto dell'uomo sui cambiamenti climatici e risposte molto significative in termini anticiclici, per sostenere la domanda, aiutare le imprese, favorire la creazione di nuovo lavoro. Il nostro dibattito poteva essere l'occasione per un passo comune verso la consapevolezza che vi sono problemi sui quali riprodurre pregiudizialmente gli steccati tra destra e sinistra non solo è insensato, ma è dannoso, tanto più che alcuni dei più impegnati protagonisti e sostenitori di uno sforzo sempre più incisivo sul fronte della lotta ai mutamenti climatici sono leader di centrodestra, come il presidente francese Sarkozy, che in una recente intervista ha detto (cito testualmente) che oggi «la sfida principale è rappresentata dal cambiamento climatico che minaccia il futuro stesso del nostro pianeta e dell'umanità intera». Poteva essere l'occasione per dare consigli utili al Governo nello sforzo anticrisi, dal piano casa all'energia, come è successo alla Camera, dove maggioranza e opposizione hanno votato insieme una mozione in cui si chiedono azioni concrete e forti per il risparmio energetico e lo sviluppo delle energie rinnovabili. Poteva essere persino l'occasione, per la maggioranza, di dare gambe un po' meno fragili e incerte ad un suo cavallo di battaglia, come l'ipotesi di ritorno al nucleare, che come unica - sia pure discutibile - giustificazione ha proprio la necessità di contribuire a ridurre le emissioni che danneggiano il clima. La discussione di oggi poteva essere tutto ciò e questi temi in effetti sono l'oggetto di molte delle mozioni presentate, come quella del Partito Democratico, ma anche quella dell'Italia dei Valori, su cui voteremo a favore, e quelle proposte dalla Lega e dall'UDC, che condividiamo largamente, su cui ci asterremo solo perché non condividiamo del tutto i passaggi sul nucleare. Poteva essere questa discussione un utile terreno di dialogo e di proposta, ma il Gruppo del PdL del Senato ha preferito imboccare un'altra strada: scrivere e forse approvarsi una mozione dai contenuti quasi surreali, che innalza la bandiera di un ridicolo negazionismo, nella quale l'allarme su questo tema e la determinazione ad occuparsene con serietà sono presentati come capricci della Commissione europea, quando sono l'oggetto di un vastissimo consenso scientifico e politico, dalla Convenzione sul clima firmata nel 1992 a Rio de Janeiro, fino alla scelta recente degli Stati Uniti di riunirsi a Copenaghen per un accordo che rafforzi ed estenda l'impegno del Protocollo Colleghi della maggioranza, se da una parte premi Nobel come Carlo Rubbia, come Steven Chu (ministro dell'energia di Obama), come Mario Molina (il chimico che scoprì l'assottigliamento della fascia di ozono e ne indicò la causa nell'uso dei CFC), insieme ai più autorevoli climatologi di tutto il mondo riuniti nell'IPCC, convengono che i mutamenti climatici in atto sono in buona parte provocati da cause artificiali, e poi qualche professore in pensione o qualche perito chimico afferma l'opposto, il risultato non è che la scienza è divisa. Sarebbe come dire che, poiché c'è qualche professore di liceo o qualche scienziato marginale che sostiene la verità scientifica del creazionismo - e in alcuni casi, sia detto per inciso, sono gli stessi che negano i mutamenti climatici - allora la scienza è divisa tra chi crede in Darwin e chi ritiene che l'uomo sia stato creato così com'è oggi. Noi voteremo contro la vostra mozione: un documento la cui approvazione non fa onore a quest'Aula e a questa istituzione. Un documento che farebbe sorridere, se mai lo leggesse, ogni serio scienziato del clima e che metterebbe in imbarazzo, se lo leggesse, qualsiasi *leader* o esponente della destra europea, o uno qualsiasi spero anche il nostro Presidente del Consiglio - dei Capi di Stato e di Governo che il 27 e 28 aprile prossimi si troveranno a Washington, invitati dal presidente Obama per concordare, come recita il comunicato ufficiale della Casa Bianca, "un impegno più forte e più incisivo per battere il riscaldamento globale". Un documento che dovrebbe far arrossire anche il Governo italiano, che ha posto la sua firma nel dicembre scorso su una risoluzione del Consiglio europeo dove si dice esattamente il contrario. Voteremo contro sperando, da italiani, che le parole strampalate della vostra mozione non indeboliscano ancora di più la già debole iniziativa del nostro Paese rispetto a un problema che segnerà la politica mondiale nei prossimi decenni e che, come ha scritto Anthony Giddens, ridisegnerà la gerarchia dei poteri e delle influenze nel mondo industrializzato, premiando chi sarà stato più pronto e lungimirante nel cogliere la necessità e l'utilità della *green revolution*.

intervengo a nome del Gruppo del Popolo della Libertà per manifestare condivisione al testo della mozione n. 107 (testo 3), in materia di cambiamenti climatici, illustrata dal senatore Possa. Caro collega Della Seta, ragionare insieme non vuole dire necessariamente darvi ragione, ma dalle sue ultime parole, che trasudano supponenza e arroganza per chi non la pensa come lei, appare invece esattamente questo. Se non vi si dà ragione, allora l'Aula non è più sovrana e, come diceva prima il collega senatore Malan, viene meno tutta la polemica che fate sull'uso degli strumenti previsti dalla norma, quale i decreti-legge. L'allarmismo che negli ultimi anni si è scatenato sul problema del riscaldamento globale, a nostro modo di vedere è esagerato. I *media* hanno capito da tempo che associare il pensiero del *global warming* a paura, terrore e disastri

hanno capito che conviene promuovere politiche sui tagli alle emissioni di CO2, perché dà loro un'ottima immagine davanti all'opinione pubblica: si tratta di un atteggiamento di omologazione opportunistica. La paura del cambiamento climatico ha da sempre colpito la fantasia dei cittadini: all'inizio del Ventesimo secolo, nel 1912, il "Los Angeles Times" titolava: «La quinta era glaciale è in arrivo: la razza umana dovrà lottare contro il freddo per salvaguardare la propria esistenza». Nessuno mette in dubbio che il clima cambi: la correlazione causa-effetto tra concentrazione di gas serra e variazioni climatiche invece non è così certa in particolare, le previsioni dei modelli basati sull'effetto serra sono poco attendibili, perché ignorano le leggi della termodinamica e perché l'«equazione clima» non è in funzione solo della temperatura, ma dell'energia complessiva che circola sul pianeta in tutte le sue forme. Evidenze sperimentali suggeriscono invece una forte correlazione tra cambiamenti climatici e attività solare. Le variazioni climatiche, nella storia del nostro pianeta, sono documentate dall'analisi stratigrafica delle successioni rocciose. La lettura di questa storia ci documenta che il clima è sempre cambiato e le variazioni climatiche sono avvenute ciclicamente con il succedersi di periodi caldi e di periodi freddi e i cicli non hanno avuto durata ed ampiezza omogenee. Le variazioni di temperatura nel corso dei tempi geologici sono state sempre accompagnate da variazioni del tenore di metano e di CO2nell'atmosfera, che hanno probabilmente ampliato gli effetti prodotti dalle cause astronomiche. le modificazioni climatiche documentate negli ultimi 2500 anni si sono succedute ciclicamente. Così le modificazioni tipo effetto serra si sono già verificate con durate di circa 150-200 anni, determinando differenti condizioni ambientali favorevoli o sfavorevoli alle attività dell'uomo nelle diverse latitudini. Il consenso scientifico sui mutamenti climatici, come ampio e privo di dubbi, esiste, con riserve, esclusivamente su tre punti. In primo luogo, la temperatura media è sempre mutevole; infatti, negli ultimi 60 anni è alternativamente aumentata e diminuita più volte e, nell'ultimo secolo, è aumentata in una misura compresa tra 0,6 e 0,15 gradi centigradi. Si è verificato, quindi, un moderato riscaldamento. La CO2, in secondo luogo, è uno dei gas serra e il suo aumento potrebbe contribuire all'aumento della temperatura;

la CO2 raddoppiasse la sua presenza nell'atmosfera provocherebbe un aumento del 2 per cento dell'effetto serra, che è dovuto principalmente al vapore acqueo e alle nubi. La terza questione sulla quale c'è consenso scientifico è che l'attività umana può essere responsabile del recente aumento della CO2, anche se molti fenomeni naturali possono causare tali aumenti. Non ci sono quindi dubbi sull'influenza dell'attività umana; noi non siamo dei negazionisti. Non ci sono dubbi sull'influenza dell'attività umana sui livelli di CO2, ma i livelli di incidenza potrebbero essere davvero limitati. Tutti gli scienziati sono però d'accordo sul fatto che anche un pieno rispetto degli accordi di Kyoto non avrebbe un impatto significativo sul clima, tenendo conto che - come dicevo prima - la CO2 rappresenta una piccola parte dell'effetto serra. Ricordo che l'applicazione integrale degli impegni di Kyoto ridurrebbe i 6 milioni di megatonnellate di CO2 prodotti all'anno a 5.850.000 megatonnellate. Capite dunque quanto poco inciderebbe. Se fossimo davvero certi della prossima catastrofe, allora dovremmo smettere di utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti fossili e tornare ad un modello di società preindustriale. Misure limitate come quelle attuali, sulle quali si fa tanta demagogia, rischiano di essere ininfluenti sul clima, ma pericolosamente dannose per il futuro della nostra economia e della nostra stessa società.

CO2. Se si tratta di definire misure anticicliche, allora possiamo considerare anche altri possibili obiettivi rispetto ai quali valutare investimenti, ad esempio l'indipendenza energetica (è stata citata oggi), o la riduzione drastica degli inquinamenti chimico‑fisici prodotti dalla combustione delle fonti fossili, che sicuramente sono dannosi per l'uomo per l'ambiente. Questi vanno ridotti e limitati. Si è a lungo discusso, inoltre, sull'inefficienza di accordi di riduzione delle emissioni di CO2 che non comprendessero gli Stati Uniti e i Paesi emergenti come la Cina o l'India. Confermando queste valutazioni, segnalo all'Aula che il disegno di legge in fase di definizione negli Stati Uniti prevede una riduzione delle emissioni del 20 per cento entro il 2020,

Peraltro, questo piano annunciato da Obama non sarà varato prima della fine del 2009, per i necessari tempi di approvazione del Congresso e del Senato, e consentirà di iniziare questa modesta riduzione non prima del 2012. Invito, quindi, i colleghi che enfatizzano questa nuova politica di Obama a leggere prima attentamente gli atti. La Cina, invece, sta mettendo in evidenza l'esigenza di considerare il consumo *pro capite* come base per definire il punto di partenza per assumere impegni sui piani di riduzione. Tale impostazione, com'è facile intuire, mette in luce la forte disparità di produzione di CO2 tra un cittadino cinese ed un cittadino occidentale. Entrambi questi Paesi, Cina e Stati Uniti, hanno dichiarato inoltre di essere indisponibili ad accordi globali vincolanti: chiedono flessibilità delle regole ed impegni esclusivamente interni, non dipendenti da trattati internazionali. Infine, da più parti si è evidenziata la funzione anticiclica, e ne parlavamo anche prima, degli investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di CO2. Vorrei dire che è anticiclico anche decidere di investire per scavare buche e per riempirle. Evidentemente è necessario scegliere misure anticicliche valutando la reale utilità degli investimenti per il presente e per il futuro ho molte perplessità che ciò lo sia, ossia la reale utilità per il futuro, per gli investimenti finalizzati a incidere in modo velleitario su presunti cambiamenti climatici legati all'attività antropica. Considerando che l'anno 2009 si prospetta come decisivo per una riconsiderazione delle politiche in materia ... *(Applausi In considerazione degli eventi internazionali che avranno luogo principalmente in Italia (G8) e a Copenaghen e apprezzata la posizione espressa dal Governo italiano nel vertice di dicembre 2008 a Bruxelles, che ha condotto il Consiglio dei Capi di Governo dell'Unione europea ad approvare una clausola di revisione da trattare nel marzo 2010 a seguito degli esiti del vertice mondiale di Copenaghen, la nostra mozione, sulla quale annuncio il voto favorevole del Gruppo, raccomanda al Governo: di mantenere la linea espressa a Bruxelles nella rinegoziazione dell'Accordo cosiddetto 20-20-20, con una minore cogenza degli obiettivi quantitativi e temporali ed evitando inasprimenti che potrebbero portare ben difficilmente credibili benefici climatici, ma certi danni per la nostra economia; di cercare accordi che coinvolgano il maggior numero di paesi emergenti; di evitare che in sede europea prevalgano atteggiamenti dogmatici, creando invece le condizioni perché prosegua il dibattito scientifico tramite il pieno coinvolgimento di quella considerevole parte del mondo scientifico portatrice di valutazioni scettiche in tema di mutamenti climatici ed antropogenici; di sostenere politiche ambientali ed anticicliche che, oltre alla riduzione della CO2 prodotta dall'attività umana concentrino gli investimenti nella ricerca di tecnologie da fonti rinnovabili e dal nucleare, che consentano la riduzione della dipendenza energetica, la riduzione degli inquinamenti chimico-fisici quali le micropolveri e le diverse sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e per la salute. Ascoltata l'illustrazione della mozione del mio Gruppo e tenuto conto del dibattito che ne è scaturito, annuncio altresì il voto favorevole del Gruppo alla mozione della Lega, di astensione alla mozione dell'UDC e contrario alle mozioni dell'Italia dei Valori e del PD. finestra"). Prima di procedere alle votazioni, avverto gli onorevoli colleghi che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

link apre una nuova finestra"). Prima di procedere alle votazioni, avverto gli onorevoli colleghi che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

Onorevoli colleghi, si è così esaurita la discussione delle mozioni sul clima. Pertanto, la seduta antimeridiana di domani è sconvocata. L'Assemblea si riunirà domani pomeriggio alle ore 15,30, anziché alle ore 16, per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni. Per quanto riguarda i lavori della prossima settimana, in relazione ai tempi di trasmissione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto‑legge "anticrisi" - il cui voto finale presso la Camera è previsto per la serata di lunedì prossimo la seduta pomeridiana del Senato di martedì 7 aprile, acquisito l'assenso dei Capigruppo, non avrà luogo. Le Commissioni chiamate ad esprimersi sul provvedimento sono fin d'ora autorizzate a convocarsi nella giornata di martedì prossimo.

e ha dichiarato incostituzionale la parte in cui si prevede l'obbligo dell'impianto di tre embrioni. Purtroppo, ci sono voluti cinque anni perché la Corte costituzionale riconoscesse che

dei bambini, perché le ha condannate a parti gemellari che comportano sempre dei rischi, sia per le madri che per i figli.

un voto che impone una legge ideologica. L'appello alla Presidenza in questo senso è che si possano finalmente trovare le modalità e l'urgenza politica per rivedere una legge che oggi la Corte costituzionale ha in parte dichiarato illegittima e incostituzionale; per riaffrontare anche nelle Aule parlamentari

fino alla giornata di ieri il Governo non ha ancora reso noti i trasferimenti erariali verso le Comunità montane, a seguito delle note modifiche legislative delle finanziarie 2008 e 2009.

esperienza di legislatore per ricordare al Governo, dall'alto delle funzione che lei oggi riveste, che l'istituto dell'interrogazione serve esattamente a questo.

non hanno lo stipendio, cioè stanno lavorando senza sapere quali soldi e da chi riceveranno dei soldi alla fine del mese, le chiedo di sollecitare con estrema urgenza una

possano o debbano ricevere lo stipendio entro la fine del mese, francamente non riesco più a capire che senso abbia il rapporto fra Parlamento e Governo. Senatore Lusi, le do atto che la sua richiesta è stata già presentata precedentemente. La Presidenza solleciterà il Governo per una tempestiva risposta